Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Liguria a seguito delle dimissioni del senatore Luigi Malabarba, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva alla quale apparteneva il predetto senatore è Adelaide Cristina Gaggio Giuliani. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Adelaide Cristina Gaggio Giuliani. Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ad una chiara pronunzia della Corte di giustizia europea, tesa ad evitare che un'imposta come l'IVA potesse alterare condizioni di parità tra gli operatori economici nell'Unione Europea, il Governo ha risposto con un decreto confuso, vago, opaco nelle modalità applicative e comunque teso ad evitare ogni obbligo. Ciò che a noi interessa è adempiere puntualmente a quella decisione nel senso favorevole ai contribuenti. Il Governo ha compiuto un'operazione assolutamente scorretta, un autentico imbroglio, perché, da un lato, ha emanato il decreto-legge n. 258 del 2006, che fa finta di dare,

per considerare l'intero periodo di imposta 2006 ben prima dell'entrata in vigore di tale decreto-legge. Riteniamo che le sentenze internazionali vadano rispettate. La vostra ambiguità è dimostrata dal non aver voluto abrogare la norma incriminata. Esponenti della maggioranza hanno messo in discussione perfino la correttezza del precedente Governo, avanzando ombre sulla linea difensiva, ponendo il sospetto di negligenze o incapacità nella presentazione di documentazioni accettabili finendo per mettere in discussione la professionalità e la competenza dell'Avvocatura generale dello Stato, in cui riponiamo piena fiducia. Un ulteriore limite è quello di aver introdotto speciali procedure senza compensazioni rispetto a quelle generali. Questo decreto non è altro che una nebbia che piomba sulle imprese, impedendo qualsiasi navigazione certa e ponendo problemi seri rispetto alla certezza dei bilanci delle imprese. È stato inoltre puntualmente disatteso il parere della Commissione politiche dell'Unione. Il Gruppo dell'UDC ha operato in senso costruttivo e propositivo, guardando alla concreta esecutività della pronuncia europea e alla creazione delle condizioni migliori per i contribuenti. Rispetto alle nostre puntuali indicazioni sono stati solo allungati i termini di scadenza per la presentazione delle istanze. È mancato ogni serio intervento che prevedesse le compensazioni fiscali, è mancata la possibilità di consentire la presentazione delle domande per via ordinaria, è mancata soprattutto la fissazione di una data certa entro la quale erogare i rimborsi. La contraddittorietà del provvedimento sta nelle confuse modalità applicative e costituisce una falsa soluzione, dimostrando la reale volontà del Governo di non dare corso alla sentenza europea, confermata dalla mancata abrogazione delle norme oggetto della censura comunitaria, e accrescendo l'indeterminatezza degli obiettivi del Governo. Questo decreto è dunque un grave imbroglio, perché, da una parte, fa finta di dare e, dall'altra, toglie con effetti retroattivi. Per queste ragioni esprimo il voto contrario dell'UDC a tale decreto, che, combinato con il decreto-legge n. 262, disattende nella sostanza la sentenza della Corte europea, viola lo Statuto del contribuente e non dà certezze ai bilanci delle imprese, sulle quali viene rigettato in modo scorretto e penalizzante il costo della sentenza.

ottimi oratori hanno evidenziato. Non mi soffermerò ulteriormente sulle discrepanze di un decreto fortemente involutivo, che consideriamo gravemente lesivo della libertà dei cittadini, delle società e soprattutto dei piccoli e medi imprenditori.

che in realtà in tutte le sue manifestazioni sta facendo evolvere un odio di classe che è più di tutto un odio rivolto contro il sistema produttivo, contro le piccole e medie imprese e contro coloro che intraprendono.

grandi sforzi in Commissione finanze e tesoro per evidenziare alcuni aspetti migliorativi, che però non ci hanno assolutamente convinto. È un decreto lesivo perché va contro gli effetti di una sentenza che comporta esborsi quantificabili in quasi 20 miliardi di euro e quindi questo adeguamento della legislazione italiana alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità dell'IVA sembra inefficace e totalmente sprovvisto nella valutazione degli oneri e della copertura finanziaria. Il provvedimento, fra l'altro, potrebbe far incorrere l'Italia in una ulteriore brutta figura e in una pronuncia europea negativa se la proposta venisse considerata meno favorevole di quella che ordinariamente disciplina i rimborsi. Non ci sorprendiamo,

una notevole frenata determinata da un eccessivo assorbimento di risorse fiscali. Il provvedimento costituisce un sostanziale aggiramento ed è in realtà, se mi passate questa

La strutturazione del provvedimento spinge a domandarsi se comporti procedure di rimborso troppo complesse, anche solo considerando l'impossibilità per il contribuente di procedere direttamente, nella fase del computo dell'IVA da versare periodicamente all'erario, alla compensazione di quanto a lui dovuto dallo Stato. Le linee del decreto comportano una forte penalizzazione dei contribuenti, ove prevedono limiti al diritto di rimborso secondo linee già bocciate in passato dalla Corte di giustizia europea. Così pure va chiarita la modalità di recupero delle detrazioni non esercitate. Tutti questi

Questo decreto viola sostanzialmente il patto di lealtà che lega lo Stato al contribuente. L'impossibilità di portare in compensazione o detrazione il rimborso spettante, ovvero l'incertezza sui tempi stessi del rimborso sostanzialmente negano i principi sanciti dallo Statuto del contribuente. Così esso vìola sostanzialmente il patto di lealtà che lega lo Stato al contribuente, ma noi sappiamo benissimo che con il Governo attualmente in carica non possiamo certamente avere patti di lealtà, perché vengono costantemente disattesi i principi reali e fondamentali della democrazia. Quindi, l'impossibilità di portare in compensazione o in detrazione il rimborso spettante, ovvero l'incertezza sui tempi stessi del rimborso non solo negano i principi sanciti dallo Statuto del contribuente, ma negano la democrazia e, soprattutto, la capacità competitiva delle nostre imprese, delle partite IVA, di tutti coloro che stanno andando avanti con grandissimi sacrifici e che verranno penalizzati profondamente e pesantemente dalla vostra finanziaria. Con convinzione il Gruppo a questo decreto-legge, non esistendo assolutamente le condizioni politiche che possano cambiare la nostra decisione e condurremo un'opposizione forte e trasparente su tutto ciò che riteniamo lesivo per il popolo italiano.

un convinto sostegno al provvedimento di conversione del decreto-legge emanato dal Governo per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella controversia che vedeva contrapposte la società Stradasfalti srl e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Trento, provvedimento che è stato ulteriormente affinato e valorizzato dall'approvazione dell'emendamento proposto della senatrice Thaler Ausserhofer, e sottoscritto anche dal nostro Gruppo, Gruppo, sia sotto il profilo di una maggiore armonizzazione del testo del provvedimento con le prescrizioni comunitarie, sia per quanto concerne il pieno rispetto dello Statuto del contribuente e la tutela degli interessi legittimi dei destinatari della facoltà di rimborso. Come molto bene hanno già esplicitato sia il presidente Benvenuto nella sua relazione all'Aula di stamattina sia i diversi interventi dei colleghi della maggioranza, il problema di fondo di questo atto deriva dalla compatibilità della normativa italiana contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il paragrafo 7 dell'articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2, in relazione alle somme versate a titolo d'imposta sul valore aggiunto negli anni 2000 e 2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli non rientranti nell'oggetto tipico dell'attività d'impresa. Quella normativa del 1972 ha poi visto nel tempo una successione di provvedimenti, posti in essere dallo Stato italiano al fine di ottenere via via la deroga, rispetto alle prescrizioni comunitarie, della disciplina vigente nell'ordinamento italiano. Ma ora, secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della VI direttiva IVA. Nel caso in cui un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stato stabilito conformemente all'articolo 17, n. 7, primo periodo, della direttiva medesima, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroghi al principio del diritto alla detrazione dell'IVA, enunciato all'articolo 17, n. 1, della stessa direttiva. Per effetto di quella pronuncia, l'IVA sostenuta sulle spese in questione è detraibile, qualora sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa ad operazioni imponibili e dell'afferenza all'esercizio dell'attività di impresa. Questa è, signor Presidente, colleghi, la situazione di fatto, rispetto alla quale appaiono sinceramente del tutto strumentali le critiche avanzate dai banchi dell'opposizione. Il Governo, infatti, ha agito doverosamente, per uniformarsi pienamente a quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia, e tempestivamente, anche per non lasciare spazi di incertezza interpretativa e mettersi in condizione di poter padroneggiare le conseguenze derivanti dall'impatto della sentenza sui conti di finanza pubblica, che non sono certo indifferenti o leggeri. Tra l'altro, ad ulteriore motivazione, sul piano tecnico si devono condurre verifiche accurate sulle singole posizioni coinvolte ed anche procedure di ricalcolo per effetti contraddittori in ragione delle imposte già versate dai contribuenti interessati da questa sentenza. Davvero, dunque, non sussistono le motivazioni a fondamento dei rilievi sollevati circa l'operato del Governo, non solo perché mi pare si sia proceduto in nome del buonsenso e della prudente ed oculata amministrazione, ma anche, e soprattutto, in considerazione della matrice da cui promana il provvedimento in questione. Perché, colleghi senatori del centro-destra, se non c'è ipocrisia, andrebbe riconosciuta quantomeno l'esistenza di un corposo profilo di concorso di responsabilità riferibile al Governo della passata legislatura. Come si evince dal paragrafo 66 delle motivazioni della sentenza e come altri hanno già richiamato, la pronuncia della Corte discende dal mancato raggiungimento di un accordo tra il Governo italiano e l'apposito comitato consultivo, previsto dalla direttiva della CEE, al quale avrebbe dovuto essere comunicata l'intenzione, da parte dell'Esecutivo che era in carica a quella data, di adottare misure nazionali in deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con quanto avvenuto, senza particolari inconvenienti, dal 1980 al 2000. Che ci sia stato errore tecnico o volontà politica, in ogni caso ciò non può esimere da un concorso di responsabilità, su cui invece l'opposizione ha disinvoltamente glissato. Anche la gestione delle conseguenze dell'impatto sui conti pubblici avrebbe dovuto trovare maggiore e più appropriato senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Stiamo parlando di cifre rilevanti, come ci ha detto il sottosegretario Grandi e come le previsioni aggiornate in DPEF e finanziaria si fanno carico di specificare. Per questo trovo contraddittorio e del tutto strumentale e preconcetto il fatto che non si sia potuto trovare un'intesa nel lavoro di Commissione sulla proposta di emendamento, poi portata all'attenzione dell'Aula, della senatrice Thaler Qui voglio dire al senatore Eufemi che, piuttosto che la debolezza della maggioranza, ciò che è risultato evidente è la chiusura e l'indisponibilità dell'opposizione. Certo, i numeri in 6a Commissione sono quelli noti, non è una novità. Ci si può annullare vicendevolmente, con discapito del lavoro parlamentare ed anche rispetto all'Assemblea; ma questa condizione potrebbe essere una bella occasione di laboratorio per un confronto di merito che valorizzi proprio il ruolo della dialettica e della progettualità parlamentare. Su questo terreno noi vogliamo caratterizzarci, com'è avvenuto anche da parte della maggioranza, sul tema in questione. La proposta della senatrice Thaler Ausserhofer cogliere il senso della discussione, di trovare un felice punto di sintesi migliorativa, consenziente il Governo, che ringrazio nella persona del sottosegretario Grandi, per migliorare il provvedimento. Nella nuova formulazione, che spero l'Aula approverà definitivamente, c'è più attenzione alla tutela dei diritti dei contribuenti; si introducono procedure più flessibili con tempi assai più ampi, come richiesto dal senatore Eufemi e in altri interventi; si facilitano le modalità di ottenimento del rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di IVA. Rigettare queste modifiche rappresenta un'oggettiva penalizzazione per la platea dei cittadini interessati pertanto un torto che il centro-destra fa ai cittadini, e non a questa maggioranza. Del resto, non penso di fare una forzatura se interpreto come un segnale di imbarazzo dell'opposizione anche la richiesta di voto disgiunto sull'emendamento approvato questa Mi rammarico che esso non sia stato chiesto in Commissione, dove evidentemente si teneva di più a marcare una contrapposizione pregiudiziale, salvo poi accorgersi, forse *a posteriori*, di essersi inflitti un vero e proprio autogol. Ne trovo conferma anche nell'atteggiamento tenuto sull'ordine del giorno approvato in Commissione all'unanimità, ma su cui, quando si è trattato di presentarlo in Aula, all'opposizione è tremata la mano.

esso interpreta proprio le preoccupazioni del centro-destra, nel senso di aprire la possibilità, in forme e modi compatibili con i saldi di finanza pubblica e con le previsioni del disegno di legge finanziaria per il 2007, di avvalersi di procedure di compensazione nei limiti e con le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Considero Considero pertanto una posizione davvero poco comprensibile, se non per sterile contrapposizione, il voto contrario dell'opposizione che, in ultima analisi, si pone come un ostacolo agli interessi di cittadini e contribuenti, che a parole, ma davvero solo a parole, millanta di voler tutelare.

Lei sa che sotto questo aspetto ho delle debolezze, quindi attenderò la collega.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questa mattina con onestà intellettuale il collega Storace ha fatto una dichiarazione di voto a favore delle dimissioni del senatore Malabarba. Ci eravamo più volte occupati in quest'Aula delle sue dimissioni, che erano state respinte certamente per la partecipazione

Con altrettanta onestà intellettuale, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale dichiaro che voteremo contro le dimissioni della senatrice Turco, non perché vogliamo continuare a confrontarci in quest'Aula con lei - questo piacere lo avremo lo stesso anche se vengono accolte le dimissioni,

dietro un voto segreto; abbiamo il dovere come senatori e a nome dei nostri rispettivi Gruppi di esprimerci in dichiarazione di voto su come ci comporteremo, in modo che questo sia fatto in maniera palmare.

le dimissioni del Ministro, nonché senatrice. Allora, noi nel segreto dell'urna voteremo contro, considerando questo come un passaggio politico. Rivolgendoci alla maggioranza, ripetiamo che i criteri devono essere uguali per tutti. Se nelle prossime ore e nei prossimi giorni apprenderemo che tutti coloro che fanno parte del Governo si dimettono da senatori,

Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà contro le dimissioni del ministro Turco. Questa mattina ho ascoltato con attenzione le motivazioni portate dalla Capogruppo di cui rispettiamo la capacità e l'intelligenza, però non riusciamo a comprendere perché quest'Aula debba essere responsabilizzata rispetto a scelte interne alla maggioranza e non capiamo neppure perché il Ministro della sanità debba dimettersi e quello della giustizia no

Sono questioni che non possono riguardare l'opposizione, trattandosi di scelte interne alla maggioranza che non possono coinvolgere responsabilità se non all'interno di una compagine che non corrisponde alla nostra.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dalla senatrice Turco. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

Lì ci sono cinque luci accese e quattro senatori; ce n'è uno che è abbastanza voluminoso, ma conta comunque per uno.